con l'esito sulla legge finanziaria, che è stata approvata da questo ramo del Parlamento. I lavori hanno riguardato, in ultimo, una lunga discussione, che ha coinvolto tutte le parti politiche, il Governo e la Presidenza del Senato, sull'introduzione nel testo di un emendamento, che era stato giudicato ammissibile parimenti ad un giudizio su altri emendamenti ordinamentali nell'altro ramo del Parlamento. Perché rimanga a verbale, ricordo che l'altro ramo del Parlamento in questo momento sta discutendo molto fattivamente su tre commi - precisamente, i commi 438, 828 e 1261 - che, introdotti con emendamento del Governo in questo ramo del Parlamento, erano invece stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza della Camera Ciò, indipendentemente da qualsiasi ragionamento rispetto all'indipendenza dei due rami del Parlamento, non può avere esito e discussione alcuna. Lo richiamo, tuttavia, perché in Commissione bilancio ci siamo comportati in maniera tale da giudicare le ammissibilità e le inammissibilità così da non far nascere questa distonia; distonia che invece è nata in modo evidente e della quale - debbo dire - nessuno si è accorto. infatti, un altro problema durante la discussione della finanziaria: la lunghezza del maxiemendamento e la gran quantità di modifiche introdotte attraverso emendamenti del relatore e del Governo non ci hanno dato la possibilità

talché il maxiemendamento non venga più riguardato e finalmente si possa varare un testo che non richieda poi decreti d'urgenza, che non richieda dibattiti, che non richieda quelle quelle accese discussioni che abbiamo visto aprirsi nelle ultime fasi dell'esame della finanziaria in questo ramo del Parlamento. Un po' più di calma, un po' più di attenzione e un po' più di rispetto del Governo per il Parlamento certamente farebbero funzionare il Senato e la Camera in modo migliore.

Signor Presidente, intervengo su una questione già posta in occasione dell'approvazione della legge finanziaria.

un errore, così com'è stato definito in una lettera inviata dal Governo alla Presidenza del Senato.

il Governo si è impegnato a comunicare per le vie brevi con quale strumento intendesse correggere tale errore, tenuto conto che la finanziaria è in approvazione alla Camera e che si esclude, per ovvi motivi, una quarta lettura al Senato. Prima

Ci dissero che non era possibile; il Governo accolse allora un ordine del giorno. L'ordine del giorno è stato poi trasformato in emendamento, condiviso in quest'Aula fra i Gruppi di maggioranza e il Governo. A questo punto, vorremmo capire dal Governo - vedo che è arrivato il sottosegretario D'Andrea

come e quando intende intervenire in materia.

che poi danno luogo a situazioni incredibili come quella che abbiamo vissuto pochi giorni fa, a deliberazioni della Giunta datate di oltre vent'anni, quando il contesto era assolutamente diverso. L'invito, è a pensare ad una strada che non passi attraverso la modifica per intanto del Regolamento, ma attraverso una disciplina di passaggi che consentano all'Aula

delle norme in esso contenute con il nostro sistema costituzionale e istituzionale. Secondo problema, Presidente, e qui mi rivolgo in particolare al Governo: che non si venga ad inserire la preannunciata norma sui reati contabili (che impedisca, cioè, l'amnistia per tali reati) in un decreto-legge *omnibus*, nel quale inserire tutto ed il contrario di tutto,

su una questione che ha riguardato la finanziaria e che ha riguardato direttamente l'Aula del Senato, peraltro, anche quando abbiamo discusso la legge comunitaria.

al presidente Marini per dire che vi era stato un errore materiale nella scrittura del comma suddetto. Il Presidente, vista l'opposizione del capogruppo Matteoli, non ha voluto aderire all'idea che fosse un puro errore materiale; noi pensiamo però che sia assolutamente necessario - e chiediamo una risposta qui, immediatamente che ci sia l'impegno del Governo alla correzione. Lo dico ancora una volta perché rimanga agli atti del Senato. Stiamo continuando a perpetuare una truffa, di cui l'Europa ci chiederà pesantemente conto, perché continuiamo a dare incentivi per cifre incredibili (come 3 miliardi) a fonti che sono tutto meno che rinnovabili, impedendo tra l'altro alle tecnologie più avanzate del nostro Paese di avere incentivi e finanziamenti. Tutto questo è pagato dagli utenti; ognuno di noi sulla propria bolletta paga ogni anno più di 60 euro per finanziare quello che non bisognerebbe finanziare. Durante l'esame della finanziaria, si era arrivati ad una soluzione a mio avviso equilibrata, equilibrata, con un testo convenuto e depositato alla Commissione bilancio del Senato. Nella scrittura del maxiemendamento vi era stato questo piccolo errore, che rende ormai la norma impossibile da applicare, che darà luogo a dei contenziosi, e chi continua a perpetuare ciò si rende complice di un danno nei confronti dello Stato. Noi chiediamo al Governo che non ci sta a sentire...

Chiti, come stanno le cose, senza impegnarsi né su come, né su quando sarà corretta la norma. Ribadiamo quindi - e io parlo a nome dei senatori Verdi e del senatore della Lista dei consumatori - che, per quanto ci riguarda, o arriva una precisazione chiara e netta da parte Governo su quale decreto opererà la correzione, oppure i senatori Verdi e della Lista consumatori non parteciperanno oggi ad alcuna votazione.

per avermi concesso la parola. Starò all'argomento introdotto dal senatore Sodano. Non parlo della finanziaria approvata, ma della questione posta dal senatore Sodano, che c'entra con la finanziaria per il futuro. Vorrei capire l'intendimento della Presidenza rispetto ad una richiesta inusuale, perché stiamo per affrontare il disegno di legge comunitaria, nella sua parte finale, e ci si viene a dire che prima di votare

non ascolta la maggioranza è un problema tra Governo e maggioranza. Proviamo però ad immaginare se le espressioni usate dal collega Sodano fossero provenute da un qualsiasi collega dell'opposizione. Si sarebbe parlato di ricatto nei confronti dei lavori parlamentari, perché si sarebbe detto che si parlava di altro rispetto al tema oggetto della discussione. Allora, Presidente, il tema oggetto della discussione non può essere riconducibile ad una specie di prova di alfabetizzazione dei Ministri, per cui commettono errori materiali nella stesura di un maxiemendamento. Infatti, ci si sta dicendo che è un ignorante il ministro Bersani che ha scritto la norma sul CIP 6,

è inaccettabile che si voglia far pensare che il Senato non si sia accorto di un errore materiale. È stata una precisa scelta politica, esattamente, come è avvenuto per quell'osceno emendamento che rischia di provocare guai

di far prestare particolare attenzione agli Uffici di Governo e del Quirinale rispetto al testo, ove mai dovesse essere approvato in Consiglio dei ministri, perché si rischia di aggiungere la beffa al danno. Cercherò di spiegarmi in pochissime parole. Vede Presidente, quest'Aula - ed è una prerogativa solo del nostro ramo del Parlamento, non dell'altro - è chiamata a pronunziarsi prima attraverso il vaglio della 1a Commissione affari costituzionali, poi attraverso il vaglio, se richiesto, dell'Assemblea di Palazzo Madama, sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di un decreto. Leggiamo - è fatto pubblico acclarato - che si sta tentando di lavorare alla modifica di questo testo, al di là della scansione temporale riguardante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che già provoca tanti problemi ai giuristi, che, se dovesse arrivare al Senato, rischia di impantanarsi sull'articolo 77 della Costituzione, in quanto stiamo parlando di un Governo che prima approfitta della fiducia, quindi imbavaglia il Parlamento, inibisce la discussione sugli emendamenti e poi lo stesso Governo dice che c'è necessità e urgenza di modificare le norme per cui abbiamo impedito al Parlamento di pronunciarsi. Credo

ma il collega Sodano e la collega De Petris**,** che si dovrebbero ascoltare quando invocano l'attenzione del Governo, hanno una possibilità: siete parte di questa maggioranza, la finanziaria è alla Camera, chiedete che si modifichino là quei commi per riportare la finanziaria qui per l'approvazione finale. Non si può fare a pezzi la Costituzione perché noi senatori dobbiamo iniziare le vacanze di Natale. Se avete forza nella vostra maggioranza, imponetela alla Camera e non piangete sul latte versato qui al Senato!

Dal punto di vista politico, non voglio mettere il dito nella piaga: è evidente che non si è trattato di uno sbaglio, ma di una scelta diversa. Non voglio entrare negli equilibri di maggioranza e chiedermi se di notte qualcuno ha cambiato il testo.

energetiche quotate e non possiamo giocare a rimpiattino su un valore nominalistico. Stiamo parlando di un evento che da stasera

sull'ordine dei lavori, per dire ai colleghi Verdi che condivido totalmente la loro battaglia, per una ragione molto politica: come Gruppo UDC, siamo stati i primi a porre la questione, ahimè senza successo, alla fine della precedente legislatura. Anche noi, infatti, riteniamo del tutto improprio prevedere vantaggi economici per aziende che, sulla base della legge, svolgono attività nell'ambito delle cosiddette fonti energetiche assimilate. Si tratta di cifre enormi che sono pagate dai consumatori

Caro Presidente, l'ordine dei lavori sta a significare che questo tema non può essere messo in discussione, né che il Governo può dire che presenterà un decreto, perché domani mattina la Camera dei deputati è sovrana e può cambiare la finanziaria. Veramente stiamo stabilendo un principio di esproprio parlamentare. Mi rendo conto che chi parte da certi espropri arriva pure all'esproprio parlamentare, ma non credo che ciò possa accadere.

(perché un termovalorizzatore costa 6-700 miliardi di vecchie lire). A tali imprese, che hanno speso

a risponderne; quelle imprese infatti si rivolgerebbero allo Stato per cercare almeno di recuperare i miliardi spesi a seguito delle autorizzazioni. La scelta del

La legge finanziaria è già stata approvata - purtroppo, dico io - da quest'Aula del Parlamento. Sono voluto intervenire per chiarire bene i termini della questione. Non si tratta di un errore materiale, ma di una scelta del Governo contraria

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, sia il senatore Manzella che il sottosegretario D'Andrea certamente non hanno bisogno di consigli e di suggerimenti, ma per registrare meglio il loro parere negli atti parlamentari, perché resti alla storia, ricordo che l'ordine del giorno è un atto che impegna il Governo,

sono stati elaborati per determinare un effetto salva-infrazione, l'uno con riferimento ai diritti consolari e l'altro con riferimento ai contratti pubblici. Sono fatti tenendo conto di alcune pronunce in corso, allo scopo di evitare il giudizio di infrazione.

seduta si era convenuto che su questo testo fosse necessario il parere della Commissione bilancio. Che questo parere fosse dato per le vie brevi o con una convocazione è un'altra questione, però non mi risulta che in Aula sia stato comunicato il parere della Commissione bilancio.

e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano perseguiti nel paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano"».

contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, che riguarda l'applicazione di una direttiva comunitaria in materia di diritto di asilo.

Quindi, i soggetti che provengono da questi Paesi (ad esempio l'Inghilterra, maestra di libertà, la Francia, maestra di libertà) non possono chiedere asilo in Italia, per il semplice motivo che la Francia e l'Inghilterra ci possono dare lezioni di libertà e di tutela

comunque concedere il diritto di asilo, se il comportamento addebitato al richiedente l'asilo è considerato in quel Paese reato e nel nostro Paese no.

quando in due Paesi, ancorché omogenei, lo stesso fatto costituisca reato o meno. Ma vi è di più. Vi faccio un esempio banale: in

uno, due o tre anni di condanna, in Italia verrebbe accolto, perché quella fattispecie non è prevista in Italia come reato. Se siamo alla commedia dell'assurdo,

dai quali l'Italia può ricevere lezioni di democrazia e libertà; in secondo luogo, se applicassimo tale norma, autorizzeremmo a chiedere l'asilo in Italia qualsiasi cittadino di un Paese sicuro

al punto di approvare una norma che chiuderà per sempre qualsiasi possibilità di controllo su chiunque voglia entrare nel nostro Paese. Cosa prevede, infatti, la norma originale?

Ricordo, ad esempio, che vi sono tantissimi Paesi africani in cui l'omosessualità è considerata un reato: basta che qualsiasi persona sbarcata

Mi dispiace che siamo arrivati a discutere ciò con il voto fondamentale di alcuni colleghi della Casa delle Libertà, che hanno garantito precedentemente il numero legale; questo mi dispiace veramente: non so

probabilmente, la mia può essere un'opinione personale, anche se non ho capito il riferimento che lei ha fatto sul numero legale, perché non mi sembrava ci fosse l'ordine dell'ostruzionismo. PRESIDENTE. Senatore, si rivolga alla Presidenza, prego. STORACE *(AN)*. È un dibattito questo, Lei avrebbe ragione - e sarei perfettamente d'accordo con il presidente Castelli - se bastasse la semplice dichiarazione dell'individuo. Nell'emendamento 12.14 (testo 4) riformulato grazie alla mediazione dell'onorevole Buttiglione, c'è scritto: «risultano perseguiti», non che dichiarino la loro tendenza, che è una cosa completamente diversa che riguarda un accertamento che viene fatto dalle nostre istituzioni. Quindi, credo che la situazione non sia così drammatica come la dipinge il senatore Castelli e dunque il mio voto sarà favorevole all'emendamento.

a titolo personale perché non ho potuto consultare il Gruppo né i membri della Commissione. Ritengo che la riflessione del senatore Castelli meriti

è da prendere in considerazione, ma è forse una differenza troppo sottile perché venga coperta e non apra, invece, con la pura e semplice dichiarazione, la possibilità dell'arrivo di personaggi che non possono essere controllati, pertanto io personalmente mi asterrò.

credo che le considerazioni fatte dal collega Castelli abbiano la loro valenza dal punto di vista di un rischio che potrebbe esserci, ma il termine che viene adoperato, «risultano», significa che l'accertamento è preventivo, vi deve essere una situazione nella quale il soggetto viene sottoposto a limitazioni di ordine penale, che in Italia non avrebbero possibilità di essere adottate. Quindi, la risultanza è preventiva rispetto a quello che sembrerebbe il passaggio libero solo sulla dichiarazione dell'interessato. Voterò dunque a favore perché mi pare che sia giusto prima di tutto preservare la differenza che separa una realtà giuridica, come la nostra, da quella di altri Paesi che hanno visioni del diritto conformi a interpretazioni puramente e semplicemente repressive.

Innanzi tutto, noi non stiamo legiferando su una norma di diretta applicazione; stiamo legiferando su un criterio direttivo e quindi c'è un'ampia discrezionalità del legislatore delegato nel conformarsi ad essa. Ma in questa conformazione è evidente che i nostri lavori costituiscono una linea secondo cui il decreto delegato potrà e dovrà essere emanato. In particolare, sottolineo cose già dette dai colleghi: in queste nostre norme, direi, le parole sono pietre. Innanzi tutto, l'insistenza sulla gravità dei motivi invocati: gravi motivi e gravi discriminazioni. Credo che il legislatore delegato non potrà sottrarsi ad una valutazione oggettiva della gravità

impegnato a porre in atto le misure necessarie ad impedire che l'esercizio del diritto sia strumentalmente usato come mezzo per evitare l'espulsione». Credo che questo nostro insieme di riflessioni debba

l'interpretazione dello stesso testo. Mi sembra che non vi sia, però, alcun dubbio che siamo di fronte ad una scelta di criterio direttivo di tipo strategico per cui diciamo che ciò che in Italia è vietato dalla legge penale è il minimo di moralità pubblica alla quale deve attenersi chi chiede asilo in Italia. Ovviamente, non bastano le dichiarazioni di chi chiede l'asilo. È un fatto preventivo, come hanno detto giustamente i colleghi Biondi e Storace. Ritengo che le preoccupazioni di un'apertura indiscriminata all'asilo in Italia vengano meno, una volta che sia chiaro che tutto ciò che è vietato dalla legge penale in Italia impedisce l'asilo politico in questo Paese, anche se esistono le ragioni di grave discriminazione. Mi sembra che questo sia un equilibrio accettabile, che apre il nostro Paese ad un asilo

di una verifica e, quindi, di un accertamento sul presupposto. Se si potesse rafforzare questo concetto con un inciso, per esempio: «risultano

unanime della norma, sia con l'eventuale rafforzativo sia con una preposizione interpretativa che, in ogni caso, toglierebbe qualunque possibilità di dubbio o di riserva da parte di alcuno.

l'estensione del diritto allo straniero, impedito nell'esercizio delle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione italiana, e quindi già tutelava un'ampia gamma

«comportamenti riferiti al richiedente e che risultano perseguiti nel paese d'origine o di provenienza». Ora, in alcuni luoghi, per il semplice fatto di appartenere a una determinata tribù, si è in qualche modo discriminati,

che viene perseguito dai regimi arabi o filoislamici, quindi, basta che uno dichiari di essere nudista. Il nudismo è un comportamento individuale gravemente represso in Arabia Saudita.

tardività di tale ordine del giorno, io mi limiterei ad accogliere la parte finale del dispositivo, che poi è la parte sostanziale: «Il Senato impegna il Governo a porre in atto le misure necessarie a impedire che l'esercizio del diritto sia strumentalmente usato come mezzo per evitare l'espulsione».

hanno partecipato colleghi di vario schieramento, sembra al Governo un punto di equilibrio soddisfacente. Quindi, siamo favorevoli all'approvazione di tale emendamento, così come risulta dal testo 4, Se l'ordine del giorno presentato dal senatore Malan si concentra

sul fatto che si sta confondendo la causa con l'effetto. Il problema non è che risultino oggettivamente o meno alcune norme o che risultino oggettivamente perseguite nel Paese d'origine alcune questioni, perché basta andare a verificare il codice penale del Paese d'origine; è chiaro che si tratta di una questione oggettiva. Il problema è che risulti oggettivamente che l'individuo che chiede asilo sia veramente perseguito per quei comportamenti. Mi spiego

bere vino; sappiamo che ciò è perseguito anche penalmente nel suo Paese d'origine. Bisognerebbe allora introdurre una norma che consenta di verificare oggettivamente il comportamento dell'individuo, non l'oggettività della norma che è evidente e che risulta patentemente *ictu* *oculi* dall'esame di qualsiasi codice penale o costituzionale. Quindi, l'aggiunta del relatore non serve assolutamente a nulla.

a me sembra singolare che comunque ci si debba impegnare a comprendere i motivi per i quali si richiede il diritto d'asilo. Quest'ultimo e le condizioni che lo rendono legittimo devono essere verificate al di fuori delle eventuali intenzioni di aggirare l'espulsione. Noi dobbiamo sempre e comunque accettare che questi elementi sussistano, indipendentemente dalle intenzioni, sulle quali non si può sindacare. Mi sembra pertanto che anche questa parte del dispositivo sia totalmente pleonastica e che finisca invece per sviare anche il contenuto della direttiva.

ringraziare i colleghi. Concordo anche perché, contrariamente a quanto alcuni colleghi hanno sostenuto, si tratta semplicemente di un emendamento di civiltà che sia la magistratura che i nostri ordinamenti

l'amarezza per un dibattito su un tema così importante che si è protratto attraverso una sorta di rateizzazione ed è arrivato in Aula

quando c'è da innovare la normativa europea e, viceversa, siamo anche i primi, i primissimi - in quei singolari sondaggi che di tanto in tanto EUROSTAT promuove

di sentirci, prima di tutto, cittadini europei, poi cittadini nazionali e, soltanto in terza istanza, cittadini delle nostre Regioni e città.

è che a questi entusiasmi ufficiali, statistici non corrispondano poi comportamenti più importanti. Siamo, come tutti sanno, i «Pierini della classe» per quanto riguarda il primato delle infrazioni comunitarie; siamo anche primi nella graduatoria, certamente non onorevole, dei richiami per quanto concerne la gestione degli aiuti di Stato, nonché per le bizzarre interpretazioni che diamo delle regole della concorrenza, che spesso pongono le Regioni in posizioni contraddittorie

dell'utilizzo e dello sfruttamento degli aiuti di Stato, soprattutto nelle Regioni dell'Obiettivo 1, che avrebbero maggiormente bisogno dei fondi a loro disposizione, ma che tuttavia, per mancanza

della Costituzione, con un gesto simbolico molto importante che riconobbe il valore dell'europeismo italiano, ma anche, consentitemi, la capacità di mediazione del Governo di allora e del presidente Berlusconi. Ora però c'è questo neo: la Costituzione non è

bizzarra discrasia che esiste in alcuni Paesi membri che magari temono, con l'applicazione di una Carta costituzionale realmente condivisa, di perdere certe *leadership* meno onorevoli; penso alla Germania ed alla Francia che hanno dettato per anni all'Europa la loro politica agricola comunitaria. Penso anche al Regno Unito, che ha fatto della mancata adesione all'Unione economica e monetaria solo l'ultima di una serie di scelte opportunistiche ispirate a quel concetto di Europa *à la carte* che sembrava superato e che, invece, ora rimane attivo e che, addirittura, viene adottato dai giovani Paesi che intendono concepire dell'Europa soltanto gli aspetti che portano vantaggi e non quelli che creano problematiche. Tutto ciò va combattuto anche in occasioni soprattutto nel settore che - lo abbiamo sentito anche poco fa in questo dibattito - è il punto nodale e critico del confronto europeo: il dominio della giustizia e degli affari interni, gli spazi di libertà, di sicurezza e di giustizia che si estendono ora verso confini comunitari sempre più vasti, in situazioni nazionali sempre meno trasparenti e più problematiche.

Esprimo un voto di astensione per questo motivo, proprio perché anche il dibattito che si è appena concluso, nonostante le aperture del relatore con cui desidero congratularmi per il difficile lavoro portato in Aula, nonostante siano Aula, nonostante siano state accolte alcune richieste provenienti da questa parte, ci sembra che il Governo non abbia ancora espresso sufficiente chiarezza e determinazione nel porre dei paletti precisi a garanzia di quelle che abbiamo manifestato come serie preoccupazioni nel settore dell'immigrazione, dell'asilo, dell'accettazione dello stato di rifugiato a fronte di mille possibili incongruenze che ancora vi sono. Questa dichiarazione di astensione è, come sempre, *double face*: un aspetto positivo riconosce una parte consistente del lavoro che è stato portato a termine, gli effetti innovativi, i segnali di adesione che dobbiamo confermare all'Unione Europea; tuttavia,

di nuovi cittadini europei, il 1° gennaio 2007 avremo una famiglia forte di 27 Paesi. Collega Manzella, quando eravamo al Parlamento europeo questa sembrava un'utopia; diciamo la verità, nessuno avrebbe scommesso su Bulgaria, e Romania, soprattutto, membri dell'Unione Europea in una data così vicina. Ora questo avviene, ma non nascondiamoci che, come per altri Paesi che entrarono nell'Unione Europea nel 2004, ciò avviene ed è avvenuto con una sorta di apertura di credito, credito, di raccomandazione sospesa che rimane per molti di questi Governi che del famoso *acquis communautaire* non erano riusciti a soddisfare tutte le voci. Se si può chiudere un occhio su determinati aspetti non fondamentali, non possiamo certo evitare di preoccuparci degli aspetti inerenti sicurezza, giustizia e libertà che condizioneranno la vita futura di tutti. Ci conforta sapere che questa materia è affidata alle mani sapienti, alla statura morale e alla capacità giuridica di un uomo come il commissario Franco Frattini, vice presidente della Commissione.

D'altra parte - come si dice - l'Europa sembra fatta, ma il popolo europeo è ancora lontano da venire. Non so se il collega Manzella ricorda il commiato di Jacques Delors nell'Aula del Parlamento europeo quando disse: non illudetevi, non esisterà mai un popolo europeo, ma popoli diversi uniti da un comune destino. Allora, rassegniamoci, nemmeno oggi costruiremo il popolo europeo, ma, credendo in questo destino, confermo l'astensione del mio Gruppo.

una materia alla quale la Lega Nord ha sempre prestato particolare attenzione. Il nostro movimento è stato l'unico ad accorgersi da subito che i commi aggiunti in sordina, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria alla Camera, non erano affatto innocui. Teniamo presente che l'impianto originale della legge comunitaria di quest'anno era già stato messo a punto dal precedente Governo e che toccava al ministro Bonino il compito di aggiungere alla lista degli atti comunitari da recepire, quelli che potevano essere stati nel frattempo imposti da Bruxelles, ed era legittimo anche introdurre criteri di recepimento, qualora la normativa comunitaria non apparisse direttamente trasponibile nel diritto interno. La direttiva è chiara, dettagliata e completa; mi riferisco alla direttiva 2005/85, che risponde a criteri di coerenza e omogeneità che il nostro movimento condivide. Ponendo criteri comuni per i rifugiati, il legislatore comunitario ha inteso anche evitare procedure illecite che, sfruttando le differenze legislative tra i Paesi europei potessero favorire illeciti. Perché allora la sinistra faziosa, che condiziona l'attuale Governo, ha imposto clausole di recepimento che vanificano il criterio di rigore o addirittura il significato della direttiva? Dalla XIV Commissione di Montecitorio è uscito un testo in base al quale se un richiedente asilo, cui fosse stata rifiutata la domanda, avesse avviato un ricorso, questi sarebbe potuto rimanere nel territorio nazionale in attesa delle decisioni del giudice, giudice, senza giustificare per quanto tempo, forse anche infinito, vista la durata media dei processi in Italia, e senza specificare a quale livello di esaurimento del processo l'*iter* potesse dirsi concluso. Praticamente una autorizzazione a oltranza e soprattutto un incentivo a presentare ricorsi, anche insensati, sempre e comunque. La Lega non poteva fare

davanti a un disposto legislativo insostenibile, irrazionale e affatto giustificabile. Trasformato il comma in un generico mandato a normare in sede di decreto legislativo la questione del ricorso giudiziario, oggi il Governo ha ammesso l'assurdità di tutto l'impianto e ha accolto i nostri emendamenti soppressivi del comma a dell'articolo 12. Resta in piedi il comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 12, che, nato a sua volta come tentativo di snaturare la direttiva, è stato prontamente contrastato dal nostro movimento fino a ridursi oggi ad un vuoto richiamo alla direttiva stessa. Ma purtroppo è arrivato l'emendamento 12.14 che, con una smodata fantasia legislativa, ha aperto le maglie sul diritto d'asilo. Avremmo preferito, signor Presidente, una norma di chiusura, non di apertura come quella proposta, una norma, questa, che non impedisce la strumentalizzazione delle disposizioni sull'asilo per permanere in clandestinità in Italia.

che fanno ricorso all'asilo quando hanno difficoltà ad avere il permesso di soggiorno. Capisco però che ci sono persone che dovrebbero ragionevolmente chiedere l'asilo e che si trovano impedite perché vengono trattate come immigrati senza permesso. Mi sembra importante in questo provvedimento proprio il tentativo di distinguere radicalmente tra asilo e immigrazione. Dunque, il Gruppo dell'UDC, che ha votato normalmente contro gli articoli della legge comunitaria,

che ci allontana dallo spirito generale di un ragionamento complessivo sull'Europa e sul ruolo che gli Stati nazionali devono avere nell'emersione delle scelte. Ma per noi che intendiamo rivendicare, non solamente l'appartenenza al nostro Partito, ma anche ad una più ampia Sinistra europea, comunque è impossibile non richiamare i temi di fondo evocati dall'argomento in discussione. L'Europa non può svilupparsi attraverso una fusione fredda, costruita su di una architettura istituzionale i cui muri portanti siano i soli parametri economici e finanziari. Se non c'è uno scatto in avanti che sia capace di rompere il velo dell'indifferenza e del sospetto di gran parte delle popolazioni che ne fanno parte, se l'Europa non è capace di suscitare attenzione ed anche un po' di amore nei suoi cittadini, questo cammino intrapreso rischia di fermarsi e di interrompersi. L'allargamento degli ambiti nazionali e l'inclusione di nuovi Paesi nell'Unione non possono trasformarsi in una diluizione del tasso di democrazia ed in una crescente distanza tra i centri di decisione ed i cittadini. Questa esigenza non è solo una nostra aspirazione, ma è leggibile anche nelle stesse difficoltà incontrate nei risultati referendari di Francia ed Olanda e nel silenzio-«dissenso» di altre Nazioni. Occorre una vera e propria cura della democrazia, signor Presidente, che dia più ruolo alle Assemblee elettive e, attraverso queste, a tutti i cittadini, a cominciare dall'apertura di una nuova fase costituente che sia centrata sul ruolo del Parlamento europeo. Signor Presidente, occorre una nuova è più incisiva politica internazionale che operi per tradurre il bisogno di sicurezza, che è tanta parte del sentire comune, non in un ripiegamento su se stessi, ma in una nuova capacità di apertura e di dialogo verso gli altri popoli e le altre culture. Occorre, ancora, che l'Europa sappia costruire e salvaguardare uno sviluppo capace di misurarsi con la necessità di mantenere in equilibrio i grandi ecosistemi, a partire dai mutamenti preoccupanti del clima. Occorre, infine, che i processi di globalizzazione ed il confronto tra i diversi sistemi di diritti e di tutele non producano un processo di svalorizzazione del lavoro quanto piuttosto la promozione di quei traguardi sociali che in questa parte del mondo i lavoratori, le loro organizzazioni ed i cittadini nel loro insieme hanno saputo conquistarsi. Èquesta una sfida che non solamente risponde ad un principio di giustizia sociale ed al dovere che abbiamo di non intaccare irreparabilmente le risorse del pianeta, ma che indica l'unica strada su cui l'Europa può recuperare e mantenere un ruolo internazionale politico ed economico, dinanzi alla tumultuosa crescita di India e Cina, mentre produrrà una ulteriore pressione competitiva sulle nostre economie, renderà inevitabilmente preziose le tecnologie e i modelli sociali ecologicamente e socialmente compatibili. Noi siamo per l'Europa dei risultati, ma solamente questi risultati possono rilanciare il progetto di una Europa dei popoli che parli non solamente per sé, ma che sia anche capace di proporre un'idea diversa dei rapporti internazionali e dei modelli di sviluppo. Sulla base di queste considerazioni e non certo spinti da una visione miope ed egoista, fondata su interessi particolari, abbiamo dato giudizi negativi sul percorso e sul punto di arrivo della Carta di Nizza abbiamo contestato la direttiva Bolkestein. Sulla base di queste considerazioni ci aspettiamo che questo Governo sappia segnare un punto di rottura, una visibile svolta, rispetto a chi lo ha preceduto. Voteremo a favore dei provvedimenti oggi in discussione anche in considerazione dei motivi di urgenza che hanno indotto ad assumere la relazione annuale relativa alla partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea già stilata dal passato Governo, accompagnandola con una risoluzione che ne ridefinisce gli obiettivi. Su questo tema, in particolare, riteniamo che dovranno realizzarsi misure più coerenti ed efficaci per perseguire gli obiettivi di Lisbona, resi difficili dalla lenta crescita economica di questi anni che, pure in un aumento quantitativo del numero degli occupati, ha conosciuto una devastante precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro. Nel confronto tra Governo e Parlamento, il disegno di legge comunitaria ha segnato significativi miglioramenti. Il ruolo dell'Assemblea elettiva ne esce rafforzato attraverso il passaggio dall'allegato A all'allegato B delle deleghe affidate al Governo per rispondere alle direttive, così come divengono più stringenti i tempi per la loro attuazione. Sul terreno delle specifiche materie, viene opportunamente introdotta una nuova delega per l'attuazione Noi, signor Presidente, ci ripromettiamo di svolgere un ulteriore ruolo nella fase successiva in cui il Governo dovrà nuovamente confrontarsi con le Commissioni e consideriamo questo di oggi un primo avanzamento verso una maggiore partecipazione delle Assemblee elettive alla fase discendente, elemento che rappresenta solo una parte del processo democratico di emersione delle scelte, un processo, certo non sufficiente, ma indispensabile alla costruzione di una Europa dei popoli e della pace, di una Europa rispettosa dell'ambiente e dei diritti delle persone, che rimane il nostro convinto ed irrinunciabile obiettivo.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, credo di potermi attribuire il merito politico di aver provocato un qualche dibattito sul disegno di perché questa discussione è cominciata in un tardo pomeriggio in cui si prevedeva di risolvere la pratica, quasi considerata fastidiosa, nel giro di un'ora.

Credo di non dover entrare nel merito della discussione perché mi sembra che si sia svolta a spizzichi e a bocconi e senza particolari linee, se non quella di fornire al Governo alcune fondamentali direttive.

di quello che può succedere o non succedere dopo il voto negativo dei popoli della Francia e dell'Olanda al Trattato costituzionale. Nei cinque anni del Governo Berlusconi si sono realizzati, con il maggiore e forte contributo dell'Italia, il più grande allargamento a dodici Paesi e, in parallelo, come conseguenza di valori euroatlantici, anche l'adesione di questi Paesi alla NATO. Sebbene ci sia stato questo duplice evento, l'Europa non ha trovato, nel campo della politica estera e della politica di difesa, una strada comune che può esservi soltanto se l'unità dell'Europa è costruita con una forte cooperazione politica e - perché non dirlo ad alta voce? - militare con gli Stati Uniti d'America. Oggi l'Occidente - intendendo, per «Occidente», valori di libertà, di democrazia, di progresso sociale, in una convivenza che noi vogliamo pacifica con tutti i popoli del mondo - si trova a dover fronteggiare il tremendo attacco (a partire da quello a New York e a Washington dell'11 settembre 2001) portato dalla «guerra terroristica», che ha come obiettivo il dominio del mondo, nel nome dichiarato di un fondamentalismo religioso e politico dell'Islam. Se l'Europa non troverà una forte unità su questi temi (ecco perché, al di là delle obbligazioni tecnico-economiche, è a questo che noi dobbiamo pensare come Parlamento, se vogliamo svolgere

ad un ordinato miglioramento delle condizioni economiche dei popoli del Medio Oriente e dell'Africa (che è il continente più vicino a noi); dove, a ragione della nostra assenza o del nostro disimpegno (soprattutto in Africa), sta crescendo l'influenza della lontanissima Cina. E per acquisire maggior respiro e maggior peso ci vogliono in Europa istituzioni valide, come previsto dal Trattato costituzionale, alla cui elaborazione il vice presidente del Consiglio del Governo Berlusconi, onorevole Fini, ha dato un apporto fondamentale, specialmente durante il semestre di presidenza dell'Italia guidata da Silvio Berlusconi. La battaglia di Fini per la citazione delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, purtroppo una battaglia perduta, non era un servizio al Vaticano, come qualche volta si è lasciato intendere, bensì il riconoscimento della storia religiosa e civile della grande maggioranza dei popoli europei. Per l'Italia le radici giudaico-cristiane hanno un significato che permane, se lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nella recente visita ufficiale a papa Benedetto XVI, ha voluto - cito testualmente - «riconoscere e apprezzare la dimensione sociale e pubblica del fatto religioso». E questa è proprio la battaglia che ha combattuto Joseph Ratzinger come cardinale, e oggi sta combattendo come Papa, perché - cito ancora - «Dio non sia espulso dalla vita pubblica». Non basta la libertà di culto, ha detto Papa Ratzinger al presidente Napolitano, la libertà religiosa è un bene più vasto. Implica il riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, secondo l'articolo 29 del Titolo II dei rapporti etico-sociali della nostra importante Costituzione italiana. Vorrei ricordare un fatto, a questo proposito; spero che il presidente Manzella, che vi ha partecipato, sia convinto di quel che dico. Sono stato negativamente stupito che, nelle settimane scorse, quando si è svolto un colloquio tenutosi su invito del Gabinetto Viesseux a Firenze, presenti il presidente Napolitano, che lo ha aperto, e il senatore Ciampi, che vi ha parlato ed ha fatto una bellissima relazione, sia mancata la voce politica di quanti al Trattato costituzionale avevano dato un apporto fondamentale, parlo in particolare di Frattini, Berlusconi e Fini, oltre che delle delegazioni parlamentari di cui facevano parte il senatore Dini e il senatore Follini, che fanno parte oggi della nostra Assemblea. Io raccolgo, di quello che è stato detto, onorevoli onorevoli colleghi senatori, quanto ha detto l'ex cancelliere tedesco, il socialdemocratico Helmut Schmidt. Ai Capi di Stato e di Governo, Schmidt ha detto in maniera chiara e coraggiosa: «Prendete le redini e ponete finalmente un freno alla burocrazia,» - senatore Manzella - «alla Commissione, ai tanti Consigli dei ministri». Nella Commissione l'Italia ora ha una garanzia politica con Franco Frattini, come l'ha avuta con Mario Monti e con Emma Bonino, due commissari che sono stati nominati

è molto di più: è una questione di eccessiva «retorica europeistica» che facciamo in Italia, con la scarsa presenza, purtroppo, non solo nella burocrazia, ma soprattutto nelle istituzioni politiche dell'Unione Europea.

l'elenco e la durata in carica dei Presidenti della Commissione europea, dalla sua nascita, nel 1958, ad oggi: nove anni al tedesco Hallstein;

Devo dire che anche nel Parlamento europeo il peso dell'Italia è scarso a causa del fatto che i *leaders* politici, quando potevano mantenere il doppio mandato, lo temevano e non andavano quasi mai a Bruxelles; oggi, invece,

Utilizzerò, quindi, da ultimo, ancora una frase, onorevole Presidente, per dire che, andando avanti in questo modo, al concetto di Europa

Quindi, è anche un lavoro comune che possiamo svolgere, in modo che alla retorica europeistica si sostituisca la concreta politica estera, economica e di difesa dell'Unione, così poco unita su temi essenziali, come lo sono quelli della libertà

senatori, normalmente l'approvazione della legge comunitaria è una sorta di atto dovuto, perché si tratta di recepire nel nostro ordinamento atti comunitari. Tuttavia, questa volta vi è un'eccessiva latitudine della discrezionalità del Governo nel recepimento e nel relativo adattamento: lo abbiamo visto in materia di articolo 12, lo vedremo anche su altri articoli. Per questo motivo dichiaro sin d'ora che esprimeremo un voto di astensione rispetto alla legge comunitaria di quest'anno. Non posso sottacere, tuttavia, che in Commissione e poi in Aula si sono ottenuti dei miglioramenti, come è il caso, ad esempio, della direttiva sui servizi finanziari, che consente un migliore coordinamento con la nuova disciplina del risparmio mentre, per quanto concerne la materia dell'asilo, è stata migliorata togliendo la lettera *b)* dell'articolo 12, anche se, tuttavia, qualche ombra continua a esserci in questa materia. È particolarmente interessante poi, soprattutto per chi si dedica alla Commissione per i rapporti con gli organismi europei, il fatto che questa legge comunitaria descriva una modalità di attuazione sia della fase ascendente sia con riferimento alle sanzioni europee, il che permetterà al Parlamento italiano di occuparsi anche di questa fase e di poter dire la propria parola in una materia così importante che riguarda il futuro del Paese non trovarsi, come spesso è successo, impreparato a recepire ciò che viene deliberato in sede europea ma poter influire anche sul processo decisionale europeo. Credo che questo non sia banale nel dare maggiore democraticità anche al sistema europeo nel suo complesso. Tuttavia, signor Presidente, non faremmo un buon lavoro se non ci ponessimo con l'occasione qualche interrogativo, soprattutto se non ci ponessimo la questione di che cosa sta accedendo all'Europa, perché stiamo attraversando una fase di ampia delusione da parte di molti nell'opinione pubblica e nei Parlamenti europei, perché in Europa i *referendum* sulla ratifica del Trattato costituzionale siano in una fase di stallo - anzi due Paesi l'hanno bocciato - e cosa succede negli altri Paesi europei e in Italia. Credo che la questione principale sia che si è voluta una costruzione europea principalmente economica, anzi monetaria, ma si è trascurata la ragione di un'Europa politica; si è perseguita un'Europa monetaria ma la conquista della moneta unica in sostanza è rimasta isolata rispetto al più ampio contesto dell'economia; si è mancato di realizzare, insieme alla moneta, o prima di essa, un vero mercato interno nel quale la moneta rappresenta, oggi come oggi, forse più un peso che non una ragione propulsiva. Questo perché sostanzialmente il mercato interno europeo risente dello schema sociale dell'Europa e non riveste le caratteristiche di un vero e proprio mercato libero e liberalizzato nel quale la competizione tra i vari Paesi e soprattutto quella tra i Paesi europei e il resto del mondo possano avvenire sostanzialmente ad armi pari. Il meccanismo complessivo delle regole europee fa sì che i Paesi europei non competano alla pari con gli altri, anzi trovino, a volte, nelle stesse istituzioni europee, dei sistemi di ulteriore complicazione, legami della loro vita. Quindi, in sostanza noi viviamo la globalizzazione non come un'opportunità ma quasi come una sorta di globalizzazione del declino che le nostre stesse regole vanno creando. Ci stiamo Ci stiamo un po' facendo male da soli e anche il meccanismo della legislazione comunitaria mostra le corde perché è francamente eccessivo; il sistema delle direttive, troppe e troppo dettagliate, finisce per rendere più difficile la vita agli europei e alle imprese europee rispetto a quelle del resto del mondo con le quali devono competere. In sostanza, non si applica non si applica un principio di sussidiarietà ma tutt'altro, si applica un principio di regolamentazione. Mentre negli Stati Uniti dal popolo si è passato alla burocrazia, sembra invece che in Europa si stia assistendo al processo inverso, cioè dalla burocrazia si cerca di passare al popolo, ma proprio i difetti di una costruzione burocratica del sistema europeo mostrano la corde e impediscono che ciò possa avvenire. Presidente, come dicevo, da un'Europa economica dovremmo passare a un'Europa politica e dovremmo, proprio per questo, cercare le ragioni del nostro stare insieme, cosa che il Trattato attuale e la Carta non hanno saputo fare perché non sono riusciti a dare un'identità vera e una voce ai cittadini europei. Se dobbiamo cercare di perseguire questo obiettivo, l'unico che dia coesione a 400 milioni di cittadini europei, dovremo costruire un vero e proprio modello culturale europeo che eviti il declino, attualmente in atto, e faccia sì che l'Europa possa tornare ad essere un faro, prima di tutto sotto il profilo culturale, anche per tanti altri popoli del mondo, che vedono nel nostro continente un modello di civiltà che andrebbe perseguito e non, invece, svilito come sta accadendo in questi frangenti.

Signor Presidente, entrambi i disegni di legge in esame sono finalizzati ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura cioè dall'UNESCO, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005. La suddetta Convenzione si propone di rappresentare la traduzione in termini normativi dei princìpi proclamati nell'ambito della Dichiarazione universale adottata in sede UNESCO nel 2001, in base alla quale il concetto di diversità culturale è elevato al rango di «patrimonio comune», inteso come l'insieme delle molteplici espressioni culturali esistenti nel tempo e nello spazio. In particolare, la Convenzione risponde a due esigenze principali: assicurare il rispetto delle identità culturali di tutti i popoli, in un contesto democratico, e contribuire all'emergere di un clima favorevole per la creatività di tutti, rendendo in questo modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile. Nel merito, la Parte I della Convenzione è dedicata alla definizione degli obiettivi, in relazione ai quali segnalo in particolare, oltre alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, l'incoraggiamento del dialogo tra culture, l'incentivo all'interculturalità, l'affermazione del legame tra cultura e sviluppo, il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati ad adottare e attuare politiche appropriate a salvaguardia del proprio patrimonio culturale e il rafforzamento della cooperazione e della solidarietà internazionale in materia. Risulta poi di particolare evidenza la Parte IV della Convenzione, la quale reca un insieme di disposizioni in tema di politiche pubbliche e misure dirette a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali e a rafforzare la cooperazione internazionale, prevedendo altresì la presentazione all'UNESCO di un rapporto quadriennale in ordine alle misure adottate sul tema in oggetto. A questo scopo si dispone che le parti aderenti istituiscano dei punti di contatto quali sedi e strumenti di ciascun Paese per la raccolta, lo scambio e la condivisione di informazioni in materia. Si tratta di strumenti dei quali l'Italia è piuttosto carente e che, al contrario, sono ritenuti essenziali per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica e dell'assegnazione di finanziamenti per le attività, la produzione e l'industria culturale. Tra i compiti assegnati alle parti contraenti figura inoltre l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale per la creazione di condizioni che conducano alla promozione della diversità delle espressioni culturali, al fine, tra l'altro, di migliorare le capacità manageriali e strategiche nelle istituzioni del settore pubblico incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica. In tema di cooperazione allo sviluppo, l'Accordo prevede una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, attraverso l'adozione di misure volte a facilitare l'accesso al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale, soprattutto per quanto concerne settori come la musica e la cinematografia, nonché mediante l'avvio di iniziative tese alla salvaguardia delle espressioni culturali a rischio di estinzione o che comunque necessitano di tutela urgente. In questo quadro, la Convenzione dispone altresì l'istituzione di un fondo internazionale per le diversità culturali, costituito per lo più da contributi volontari degli Stati membri, il cui utilizzo sarà stabilito dal Comitato intergovernativo, sulla base di linee guida determinate dalla Conferenza degli Stati aderenti. L'accordo prevede inoltre l'istituzione di una Conferenza degli Stati aderenti, la quale si riunisce una volta ogni due anni per eleggere i membri del Comitato intergovernativo, approvare le linee guida operative della Convenzione

ringrazio, Presidente. Il Comitato intergovemativo si riunisce invece annualmente e definisce le linee guida per l'attuazione della Convenzione, promuove gli obiettivi della Convenzione e svolge il monitoraggio sull'attuazione della medesima. È inoltre previsto che l'assistenza agli organi della Convenzione sia garantita dal Segretariato dell'UNESCO. Un'attenzione specifica è infine dedicata ai rapporti con le organizzazioni regionali di integrazione economica, con riguardo al caso specifico dell'Unione Europea, che prelude all'adesione della stessa Unione (una (una volta che a questa verrà conferita personalità giuridica o nel frattempo alla Comunità economica europea), che si affiancherà alle ratifiche degli Stati membri. Al riguardo, nell'accordo si chiarisce che i diritti previsti dalla Convenzione non saranno esercitati cumulativamente, bensì alternativamente, o dall'Unione, in ragione del coinvolgimento di competenze comunitarie riguardanti i profili inerenti agli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, o dagli Stati membri; laddove sia l'organismo europeo ad esercitare i diritti di voto, esso disporrà di un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti della Convenzione. Tali specifiche procedure di adesione evidenziano l'eccezionalità di questo testo convenzionale nel panorama delle iniziative negoziali dell'UNESCO, che mai prima aveva sperimentato la diretta partecipazione dell'Unione Europea ai propri lavori. La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, signor Presidente, appare pertanto coerente sia con il tradizionale impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, sia nel quadro UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT), sia con lo specifico contributo dato all'adozione della Convenzione in argomento, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo. Signor Presidente,quanto al testo del disegno di legge n. 890, d'iniziativa della senatrice Vittoria Franco ed altri, si rileva il carattere sostanzialmente identico a quello del Governo, il disegno di legge n. 1179, salvo che quest'ultimo reca le necessarie disposizioni di copertura finanziaria. Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione affari esteri ha ritenuto di adottare come testo base il disegno di legge n. 1179 e ha conferito mandato

Signor Presidente, la Convenzione sulla diversità culturale e delle espressioni artistiche dell'UNESCO, che oggi ci apprestiamo a ratificare, venne definita, al tempo della sua adozione, dopo tre difficili anni di negoziati e dibattiti, come una prima ma importante vittoria morale nella lunga via per la protezione della ricchezza e diversità culturale del pianeta. In molti allora definirono la Convenzione, adottata a stragrande maggioranza con il solo voto contrario degli Stati Uniti e di Israele, una vittoria dell'Europa e della sua determinazione a proteggere e promuovere la propria arte e cultura nei confronti della cultura di massa statunitense, la cosiddetta cultura di Hollywood. C'è un precedente importante che vale oggi la pena di ricordare ed è il fallimento a suo tempo del negoziato sull'accordo multilaterale sugli investimenti, il cosiddetto MAI, che si arenò proprio sull'indisponibilità della Francia e di altri Paesi europei a rinunciare alla cosiddetta clausola di salvaguardia culturale, osteggiata invece dagli Stati Uniti che avrebbero preferito una completa liberalizzazione del mercato dell'arte, della cultura e degli audiovisivi. Questo fattore oggi viene capovolto dalla Convenzione UNESCO. Cultura e Arte vengono finalmente definiti come bene comune indisponibile alle leggi del mercato, e viene riconfermato un approccio multilaterale e «pattizio» come strumento di garanzia di tutela di tale bene comune. In un certo senso la Convenzione si pone come primo vero strumento di «governo» della società multiculturale, riconoscendo la centralità della diversità e delle varie forme di espressione culturale e artistica, compiendo un importante passo in avanti per il superamento del relativismo culturale. Restano alcune questioni irrisolte, a nostro parere, prima fra tutte la compatibilità di questa Convenzione nei confronti delle regole delle liberalizzazioni del commercio, le cosiddette regole GATS sui servizi del WTO e quelle per i diritti di proprietà intellettuale. Restano anche le preoccupazioni rispetto all'iniziativa che l'Unione Europea sta svolgendo di inserire la liberalizzazione dei servizi, e quindi anche il settore culturale e audiovisivo, come una delle condizioni da porre negli accordi bilaterali commerciali con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (i cosiddetti accordi di partenariato economico). riteniamo che l'Italia oggi, facendo questo primo passo verso la ratifica della Convenzione UNESCO, debba anche rappresentare in tutte le sedi, soprattutto quelle commerciali e verso i Paesi in via di sviluppo, la centralità del diritto alla cultura come bene comune e l'indisponibilità della produzione culturale e artistica alle leggi del mercato e del libero investimento. Vorrei concludere ricordando che la Convenzione è stata frutto di un'importante interazione critica tra Governi e società civile: questa deve essere mantenuta anche nel processo di implementazione a livello nazionale. I punti di cultura e di contatto devono quindi essere aperti anche alle proposte e ai suggerimenti della società civile organizzata nel nostro Paese.

Presidente, come Governo ci eravamo riservati di fare questa precisazione. Del resto, è già stato emesso un comunicato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha confermato la posizione già assunta dall'Esecutivo in questa sede. prossimo si svolgerà un'apposita riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio, con la partecipazione dei Ministri interessati, nel corso della quale saranno definite le modalità con cui, nei giorni immediatamente successivi, saranno apportate al provvedimento le correzioni in materia di CIP 6, nel senso più volte dichiarato in quest'Aula e

gravi. Il Governo, infatti, ha detto di voler ribadire la posizione espressa attraverso un comunicato della Presidenza del Consiglio che, a sua volta, avrebbe confermato la posizione qui espressa dal Governo sulla questione legata ai rifiuti, che è quella contenuta nel maxiemendamento alla finanziaria su cui ha imposto la fiducia. Non vi è stata qui altra posizione del Governo, Presidente; non si può allora venire a gabbare, peraltro in questo periodo, nel momento in cui alla Camera dei deputati è in discussione la finanziaria. Tali comunicazioni sono irricevibili. Il Governo ha il dovere, se crede di aver commesso un errore nella stesura del maxiemendamento, di andare alla Camera e presentare un emendamento correttivo; pensare, dopo aver imposto la fiducia al Parlamento, di emanare un decreto per correggere non un errore materiale, ma una scelta politica non si giustificherebbe per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e sarebbe molto grave la quiescenza della stessa Presidenza del Senato di fronte a questa prepotenza.

comunica che le Commissioni potranno convocarsi a partire dal 15 gennaio 2007, giorno in cui riprenderanno dunque i lavori del Senato della Repubblica. Ove lo ritenessero opportuno, peraltro, le Commissioni medesime potranno convocarsi sin da martedì 9 gennaio. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 23 gennaio, alle ore 17, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La Conferenza dei Capigruppo sarà preventivamente convocata per la definizione del calendario nei giorni successivi. Cari colleghi e colleghi, rivolgo a tutti voi, anche a nome del presidente Marini e dell'intero Consiglio di Presidenza, i più vivi e fervidi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Colgo l'occasione per rivolgerli anche alle vostre famiglie.

ringrazio e buone festività a tutti.

necessario l'intervento delle forze dell'ordine. C'è un interessamento del prefetto di Roma; c'è una situazione di emergenza per la quale il sindaco di Roma, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione hanno chiesto la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, sarebbe necessario un intervento del Ministro dell'interno a garanzia di una zona importante dell'estrema periferia romana.